Mi riferisco all'interrogazione del senatore Zanda con la quale chiede informazioni in merito alle dimissioni dei membri italiani del Comitato scientifico del Musée du Luxembourg. Al riguardo vorrei preliminarmente evidenziare che l'organizzazione delle mostre sull'arte italiana al Musée du Luxembourg è stata sino all'estate del 2008 il frutto di un meccanismo basato sulla collaborazione tra la responsabile artistica del museo per le mostre sul Rinascimento italiano, Patrizia Nitti, e il Comitato scientifico di cui erano membri, a titolo personale, gli esperti e curatori del nostro patrimonio menzionati nell'interrogazione. Il predetto meccanismo è saltato in seguito ai contrasti sorti tra la signora Nitti e il titolare della società di gestione del museo, Sylvestre Verger. La decisione dei cinque membri italiani del Comitato scientifico di rassegnare le dimissioni trova infatti le sue ragioni - come spiegato dagli stessi dimissionari in una comunicazione al museo nel venir meno della situazione che aveva consentito fino a quel momento di operare in un clima di serenità e fiducia reciproca (sostanzialmente a causa delle crescenti pretese del Verger di ampliare il suo ruolo e dell'allontanamento della signora Nitti). L'azione del Ministero per i beni e le attività culturali, non direttamente coinvolto nel descritto meccanismo, si estrinsecava in concreto nell'autorizzare la concessione in prestito delle opere d'arte a fronte dei progetti espositivi presentati dal predetto Comitato scientifico e dei pareri favorevoli espressi dalle soprintendenze competenti. Per tali ragioni, una prestigiosa mostra sui Medici, prevista per il 2008-2009, non ha più è stato peraltro sostituito nel novembre 2008 per raggiunti limiti di età da Gérard Larcher. Quest'ultimo ha disposto immediatamente un'indagine sul funzionamento del Senato, ivi inclusa la gestione del Musée du Luxembourg, da concludersi entro il mese di giugno 2009. Nel frattempo, pur in assenza di un Comitato scientifico funzionante, il museo ha ha organizzato una mostra su Filippo e Filippino Lippi, di cui il nuovo presidente Larcher si è assunto la piena responsabilità e in relazione alla quale la soprintendenza di Firenze ha espresso un parere favorevole alla concessione in prestito delle opere d'arte. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha eccezionalmente autorizzato il prestito delle suddette opere d'arte, in un'ottica di buone relazioni con il Senato francese e al fine di dimostrare concretamente al nuovo Presidente il desiderio di veder ripristinate le condizioni di una serena collaborazione per la realizzazione di mostre prestigiose. Da ultimo, sulla base delle risultanze della summenzionata indagine concernente il funzionamento del Senato, il 1° luglio scorso il presidente Larcher ha annunciato

al termine della prossima esposizione già messa in cantiere sulla gioielleria Tiffany, la cui chiusura è prevista nel gennaio 2010). Pertanto, al posto dell'attuale "autorizzazione d'occupazione temporanea" - come viene tecnicamente definita la relazione con il Verger - verrà istituita una "delegazione di servizio pubblico", meccanismo più consono alla natura pubblicistica del Senato. Data la necessità di una sorta di gara d'appalto, è presumibile che si dovrà attendere un certo lasso di tempo prima che la nuova struttura cominci ad essere operativa. Solo a quel Solo a quel momento sarà possibile verificare l'opportunità o meno di autorizzare la concessione in prestito di opere d'arte per future mostre organizzate presso il Musée du Luxembourg. Vorrei inoltre rappresentare al senatore Zanda che l'autorizzazione al prestito delle opere d'arte viene rilasciata dal Ministero attraverso la competente direzione generale nella stretta osservanza del combinato disposto degli articoli 48 e 66 del codice dei beni culturali e del decreto ministeriale 29 gennaio 2008, recante le linee guida elaborate dall'apposita commissione ministeriale istituita con decreto ministeriale 5 settembre 2006 che ha, fra l'altro, sancito i seguenti principi in materia di attività di scambio, prestito e collaborazione tra istituti museali e altre istituzioni culturali: il principio di normalità, nel senso che la predetta attività va considerata ordinaria e finalizzata all'accrescimento della della qualità dell'offerta culturale nel suo complesso; il principio di sostenibilità, in modo che il beneficio netto per il sistema culturale ne risulti positivo; il principio di qualità, perché il prestito deve essere subordinato all'accertamento della coerenza e della qualità culturale della manifestazione per la quale è richiesto, giustificando la rinuncia temporanea all'opera stessa in nome di un avanzamento culturale; infine il principio di ricaduta, perché il prestito deve essere subordinato all'accertamento del ventaglio di benefici materiali, immateriali, culturali e identitari, che derivano all'istituto proprietario, al suo territorio e al Paese, dall'inclusione dell'opera nella mostra. Preciso, infine, che il procedimento autorizzatorio prevede una istruttoria di merito svolta dalla predetta direzione generale a partire dal parere favorevole espresso dalle sopraintendenze competenti che garantiscono, oltre allo stato di conservazione delle opere, la qualità culturale dei progetti espositivi e la sicurezza delle medesime nelle fasi del trasporto e dell'esposizione. Viene, inoltre, acquisito il parere conclusivo, ove previsto, dell'apposito Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *c*), del decreto del organo consultivo della citata direzione generale.

Sottosegretario anche per la completezza della risposta e rubo pochi minuti all'Aula per indicare alcuni elementi di insoddisfazione riguardano, oltre che il tema specifico dei nostri rapporti con il Musée du Luxembourg, la politica del nostro Paese in particolare del Ministero per i beni culturali rispetto al tema delicatissimo del prestito delle opere d'arte per l'organizzazione di mostre. Riguardo al tema specifico del museo, signor Sottosegretario, devo rilevare la

Davanti a questo *deficit* di garanzia culturale io avrei posto maggiore attenzione nel proseguire la collaborazione che ha prodotto la mostra su Filippo Lippi.

abbiamo ascoltato dalle sue parole, in modo ripetuto, la necessità di espletare gare corrette, abbiamo sentito parlare di appalti, abbiamo udito di contrasti tra la cultura e gli elementi culturali di un museo e i responsabili della gestione. Ebbene, credo che

il rapporto generale che deve avere lo Stato italiano con chi organizza le mostre all'estero ed anche nel nostro Paese. Mi sembra che nel nostro Paese sia eccessivamente diffusa la moda di organizzare grandi mostre d'arte soltanto per motivi commerciali. Ritengo che ci sia un eccesso di discrezionalità nel giudicare il valore culturale di una mostra.

straordinarie opere d'arte, ma anche una parte consistente dell'immagine dell'Italia alla quale il suo Governo, l'Esecutivo di cui lei fa parte, tiene tanto. parte, tiene tanto. L'invito pressante che le faccio in questa sede è di esprimere un indirizzo chiaro, se possibile tornando in Parlamento per comunicarci qual è veramente il criterio di fondo con con cui il Governo intende procedere in questa materia, quali regole intende seguire e come intende farle osservare a partire, naturalmente, dal personale personale del Ministero e delle sovrintendenze, la cui qualificazione scientifica non è assolutamente in discussione. Quando però si tratta di organizzare mostre d'arte abbiamo

datato 9 febbraio 2007, con il quale veniva ordinata la predetta rimessione in pristino, è stato oggetto di ricorso giurisdizionale con il quale i comproprietari dell'immobile ne chiedevano l'annullamento, ritenendo la porzione immobiliare di loro proprietà non interessata al vincolo monumentale

ha definitivamente respinto il ricorso in appello avanzato dai comproprietari per l'annullamento della precedente sentenza n. 3637 del 2007 pronunciata dal TAR Veneto che, già in primo grado, non aveva accolto l'impugnativa dei ricorrenti. Successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato, la soprintendenza per i beni architettonici di Venezia ha autorizzato l'esecuzione di una campagna di indagini tecniche e statiche ai sensi dell'articolo 21 del codice dei beni culturali, volte a verificare la fattibilità edilizia del ripristino dei dei luoghi presso Palazzo Zabarella. A tal proposito, voglio rassicurare il senatore interrogante circa il fatto che le predette indagini non sono volte ad eludere il decreto di rimessione in pristino in questione, ma sono anzi propedeutiche all'esecuzione dello stesso. Il decreto, infatti, dispone, fra l'altro, che la rimessa in pristino dello stato dei luoghi avvenga anche "dell'accurata rimozione, previa esecuzione dei saggi conoscitivi e testper accertare la consistenza delle strutture che sostengono il pavimento della terrazza, di tutte le opere eseguite in assenza di autorizzazione..." e con e con le esigenze di tutela monumentale dell'immobile in questione. Voglio pertanto confermare l'impegno di questo Ministero per dare piena e concreta esecuzione al citato provvedimento di rimessione in pristino, anche attraverso il preliminare svolgimento delle suddette attività di indagine, finalizzate esclusivamente all'individuazione di idonei interventi per la salvaguardia dell'integrità di Palazzo Zabarella.

delle Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso sembrava avere alcune parti in contraddizione rispetto a tutti gli altri provvedimenti, da quello del Consiglio di Stato

rispetto alla tutela della cultura e del patrimonio artistico, debba fare in modo che quel patrimonio straordinario, consegnatoci da generazioni di persone, non solo venga tutelato, ma rimanga e venga consegnato al futuro. Se viene meno questo impegno, oppure - come le ho richiamato nella lettera del 9 febbraio 2009 - esso è perlomeno sottaciuto, rallentato, c'è il rischio che questo patrimonio subisca dei danni. ci darà atto che almeno da parte dell'opposizioni in questo caso, non in maniera gridata, l'aver presentato questa interrogazione, l'averla sollecitata più volte in Commissione, vuol dire che nutriamo gratitudine e profondo rispetto verso quei privati che anche con sforzi economici tutelano patrimoni artistici importanti. Sappiamo però anche che vi sono interessi superiori, come la tutela del nostro grande patrimonio artistico, che lo Stato deve garantire sopra ogni cosa, con l'autorevolezza necessaria.

perché ci sembra un dato di rispetto della proprietà legittima ed anche un dato di rispetto di quanti hanno a cuore l'arte di quella città, che è poi un patrimonio di tutto questo Paese.

con riferimento all'interrogazione del senatore Vita con la quale chiede di conoscere le valutazioni del Ministro in ordine alla riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alle nuove nomine dirigenziali e, segnatamente, a quelle esterne al personale in organico al Ministero, faccio presente che il decreto del Presidente della Repubblica del 2 luglio 2009, n. 91, ha ridefinito la struttura organizzativa degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali. A norma dell'articolo 2, comma 7, dello stesso decreto, la suddetta riorganizzazione ha dato luogo alla revoca anticipata degli incarichi dirigenziali in corso, per motivate ragioni organizzative e gestionali, in applicazione di quanto previsto dall'art. 20,

ha previsto la sostanziale innovazione delle strutture dirigenziali di livello generale, in particolare per quanto concerne le missioni istituzionali, e la rivisitazione delle competenze alle stesse attribuite, a livello centrale e periferico. Le modificazioni apportate sono state tali da rendere necessaria la ridefìnizione dell'oggetto di tutti gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale in atto e degli obiettivi agli stessi connessi, al fine di renderli coerenti con i nuovi poteri di coordinamento e gestionali attribuiti ai responsabili delle singole strutture. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha correttamente operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che regolano la materia del conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale. Infatti con circolare n. 205 del 20 luglio 2009, la competente direzione generale per l'organizzazione, la formazione, l'innovazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali ha comunicato la disponibilità degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 16 maggio 2007 con il quale sono dettati i criteri per l'attribuzione di detti incarichi. L'Amministrazione ha pertanto proceduto all'esame ed alla valutazione delle richieste di conferimento degli incarichi dirigenziali, tenendo presente l'interesse pubblico prioritario di individuare il dirigente avente le competenze professionali e le capacità manageriali più idonee a garantire l'ottimale ed efficace svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi, nonché le preferenze manifestate, tenendo comunque conto dell'esigenza di assicurare il buon andamento e la piena funzionalità dell'amministrazione. A tal fine, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi connessi agli incarichi, si è tenuto conto delle peculiari attitudini, della comprovata esperienza, della particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica e delle capacità manageriali dimostrate nello svolgimento di precedenti incarichi o attività. Sulla base di una articolata valutazione comparativa delle istanze prodotte e dei relativi *curricula*, sono stati individuati i soggetti più idonei a ricoprire gli incarichi di direzione delle strutture centrali e periferiche. Per quanto concerne poi gli incarichi conferiti al personale estraneo all'Amministrazione, ed in particolare quello di responsabile della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, determinanti nella scelta del nuovo direttore generale sono state le notevoli competenze ed esperienze professionali, nonché le ottime capacità manageriali dimostrate in precedenti qualificate esperienze di lavoro nell'ambito della imprenditoria privata. È stato fondamentale, inoltre, per questa Amministrazione avvalersi, in una materia di rilevanza strategica quale quella della valorizzazione del patrimonio culturale, di una risorsa umana dotata di alta professionalità e di accertata esperienza manageriale, come ampiamente documentato dal *curriculum vitae* del prescelto. Circa poi agli spostamenti di personale dirigenziale in sedi non indicate nelle preferenze manifestate, si fa presente che tale circostanza si è verificata in misura molto contenuta ed ha trovato comunque fondamento, come sopra chiarito, nella prioritaria prioritaria esigenza di assicurare la funzionalità ed il buon andamento dell'amministrazione su tutto il territorio, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che regolano il conferimento degli incarichi dirigenziali ed il trattamento giuridico ed economico dei dirigenti. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Giro per le parole che ha voluto usare, pacate e anche molto formali, certo frutto di qualche generosa - immagino - di un ufficio legislativo: so per esperienza che spesso così accade, nella sottovalutazione che in generale i Governi hanno dell'opera ispettiva dei parlamentari. Signor Sottosegretario, l'interrogazione da me presentata ha un senso molto preciso: tende a porre con allarme l'attenzione sulla discrasia tra le attese di un Paese che vive fondamentalmente grazie al suo patrimonio culturale - così è

diverse osservazioni critiche che l'opposizione svolse su quel decreto da lei evocato *ab origine* della sua risposta come cemento della medesima. Si pone

Ci sono a volte degli specialismi rigorosamente necessari, quella passione che viene da una dedica antica, come dicono alcuni grandi maestri di musica: ci sono alcune attività della vita artistica che non si possono apprendere ad un certo punto, quando si è troppo adulti, perché bisogna aver amato queste cose da piccoli per poter dedicare la propria vita ad una straordinaria opportunità per l'Italia. La seconda questione forse si potrebbe trovare un termine italiano. Perché alcuni direttori sono stati spostati? È stata tra l'altro abolita la direzione PARC, molto buona in verità

che quanto è accaduto con la riorganizzazione del Ministero non solo è andato oltre lo spirito stesso del decreto da lei evocato, ma ha messo in moto qualcosa che poi lo stesso nostro

con riferimento all'interrogazione del senatore Andria concernente la riorganizzazione degli uffici dirigenziali periferici del Ministero, con particolare riguardo agli uffici con sede a Salerno, faccio presente che con decreto ministeriale del 20 luglio 2009, concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state confermate sia la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggisti per le Province di Salerno ed Avellino, sia la Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici per le medesime Province. Circa la richiesta di riconsiderare il ridimensionamento degli uffici periferici di questo Ministero, rappresento che l'Amministrazione ha dato attuazione e seguito ai criteri previsti dal disposto normativo previsto dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,

per effetto dell'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). La riduzione da ultimo operata incide a livello centrale con una percentuale di circa il 17 per cento e a livello periferico con la percentuale di circa l'8 Ciò al fine di mantenere il più possibile la presenza sul territorio degli uffici con competenze tecniche, che svolgono le rilevanti funzioni di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Desidero però soffermarmi per qualche attimo sulle questioni a monte che dettarono in me la necessità di ricorrere ad un'interrogazione rivolta al Ministro per i beni e le attività culturali. Bisogna considerare il contesto territoriale al quale mi riferisco affinché possa essere compresa fino in fondo la preoccupazione di cui mi resi interprete attraverso l'interrogazione di cui ci si occupa, allorché si diffusero notizie veramente allarmanti circa l'ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero per i beni

Sono due le considerazioni a monte da fare: la forte concentrazione di patrimonio culturale e storico‑artistico in entrambe le Province e, naturalmente, l'altrettanto forte concentrazione di patrimonio ambientale e paesaggistico. Basti pensare che la Provincia di Salerno, tra le due, è quella che recentemente, qualche anno fa, è stata toccata da interessanti ed utili provvedimenti quando ha ottenuto, nella lista UNESCO del patrimonio mondiale dell'umanità, prima l'iscrizione della costiera amalfitana e successivamente del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con alcune emergenze architettoniche e archeologiche che insistono in quel territorio. Appare chiaro che, nel caso in cui quelle notizie, che in quel momento ‑ parlo delle prime settimane di maggio ‑ erano piuttosto ricorrenti, avessero trovato rispondenza, il territorio delle due Province di Salerno e di Avellino ne sarebbe stato veramente turbato, avrebbe subito una deprivazione di strutture di straordinaria utilità per la tutela e la salvaguarda del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico‑artistico.

‑ naturalmente mi riferisco al personale ‑ sarebbe andato disperso e sarebbe stato non sufficientemente utilizzato. Ricordo a me stesso che l'ipotesi che si paventava era quella di un accentramento dei compiti direzionali

invece, regolarmente quella per i beni ambientali e paesaggistici. Parlo di funzionamento non del tutto regolare perché nella Soprintendenza ‑ approfitto della presenza del signor Sottosegretario per segnalare questa situazione

dunque, c'è una difficoltà. Occorre che il Ministero, signor Sottosegretario, si attivi presso il direttore regionale della Campania al riguardo.

‑ alla gestione del personale devono appoggiarsi alla Soprintendenza per i beni ambientali e paesaggistici. In conclusione, nel ribadire la mia soddisfazione per la risposta che in Aula il Sottosegretario ha reso a nome del Governo, segnalo con l'occasione alla sua attenzione, signor Sottosegretario, la necessità di disporre con tempestività in ordine alla nomina del soprintendente ai beni artistici e storici, nonché alla definizione della pianta organica della medesima Soprintendenza. la vicenda del medicinale Ubidex risale al 2002, anno in cui fu effettuata un'ispezione ministeriale presso l'Officina farmaceutica fiorentina dalla quale emersero 119 deviazioni, a seguito delle quali l'Officina è stata sospesa. Successivamente all'intervento del Comando dei carabinieri per la tutela della salute, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il 23 aprile 2008 ha emesso un provvedimento di ritiro e di divieto di vendita di tutti i medicinali prodotti presso l'Officina suddetta. Poiché l'Azienda ha ottemperato solo in parte alle procedure di ritiro, a maggio 2008 i NAS hanno diramato le disposizioni di sequestro sul territorio nazionale di tutti i medicinali di cui la ditta OFF srl. risultava essere titolare di autorizzazioni al commercio. A seguito della richiesta presentata dall'Azienda per il rinnovo dell'autorizzazione al commercio per l'Ubidex, l'AIFA ha comunicato che tale rinnovo non poteva essere rilasciato, in quanto l'Azienda non è stata in grado di esibire un documento attestante l'autorizzazione a produrre da parte di un'officina, né ha presentato una richiesta di variazione per la sostituzione dell'officina di produzione revocata. Inoltre, non è stato fornito alcun riferimento valido per la certificazione di *Good Manufacturing Practice* (GMP) del produttore della sostanza attiva, né alcuna dichiarazione, a firma della *qualified person*, attestante la conformità alla GMP, né il piano

dell'autorizzazione al commercio della specialità medicinale Ubidex-50 milligrammi capsule (provvedimento del 14 novembre 2008 confermato con determinazione del 30 giugno 2009). L'AIFA ha, peraltro, precisato di non aver ricevuto tramite la Rete nazionale di farmacovigilanza segnalazioni di reazioni avverse associate all'assunzione di questo medicinale. Relativamente alla Regione Sardegna, l'ente regionale ha precisato che le ASL di Sassari, Nuoro, Oristano, Sanluri e Carbonia non hanno mai acquistato, né dispensato l'Ubidex. Soltanto le aziende sanitarie locali di Olbia e Cagliari hanno dispensato il prodotto fino all'aprile 2008. L'ASL di Olbia ha provveduto al ritiro immediato del medicinale a seguito del citato provvedimento dell'AIFA. L'ASL di Cagliari aveva acquistato 350 confezioni di Ubidex nel 2007 e 56 nel 2008, dispensandole a cinque pazienti con patologie cardiache e non, A seguito delle segnalazioni pervenute al Servizio farmaceutico della ASL suddetta, che evidenziavano anomalie di confezionamento e che sono state debitamente comunicate all'AIFA, per i lotti difettosi è stato disposto il ritiro su tutto il territorio nazionale con provvedimento dell'AIFA del 10 aprile 2008. L'ASL ha immediatamente sospeso la relativa fornitura ai pazienti in trattamento, disponendo la sostituzione del farmaco con altre specialità a base di ubidecarenone. I medicinali non utilizzati sono stati sequestrati dai NAS presso l'ASL di Cagliari il 28 maggio 2008. In merito ai dati sulle confezioni vendute dall'anno 2002 al 2008 è a disposizione la relativa tabella, con la precisazione che il dato per il 2008 è riferito solo al primo trimestre, in quanto nessuna confezione risulta venduta nei rimanenti tre trimestri. Signor Presidente, ringrazio il signor Sottosegretario per la risposta che ha voluto dare in quest'Aula.

questa intimazione, che ha il suo peso e la sua forza legale, sia rimasta disattesa. Questo non può e non deve accadere. Devono esserci i mezzi coercitivi per impedire

balia di questi malfattori quando non mi pare che possiamo consentire una cosa del genere, soprattutto in un settore così delicato che riguarda la salute dei cittadini, tutelata dalla Costituzione repubblicana. Le affido pertanto il compito di riferire al Ministro

fatto affidati ad autorità competenti che devono fare il loro dovere, dai NAS all'Arma dei carabinieri in generale, dalle ASL agli uffici di Polizia. Occorre fare tutto quello che è possibile per impedire queste gravissime illegalità nella commercializzazione di prodotti fantasma. Parliamo tanto di quelli che arrivano dalla Cina, ma ci sono anche quelli prodotti in Italia; dunque, non ci scandalizziamo più di tanto gridando sempre "al lupo, al lupo" nei confronti degli altri, ma guardiamo prima casa nostra e facciamo il nostro dovere.